Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche al calendario corrente dei lavori dell’Assemblea. In relazione all’andamento delle Commissioni riunite 1ª e 5ª, l’avvio della discussione del decreto-legge in materia di proroga termini, giaprevisto per la seduta odierna, e stato rinviato alla giornata di lunedı14 febbraio, con inizio alle ore 16,30. Le Commissioni proseguiranno i loro lavori nella giornata odierna e anche nei prossimi giorni, al fine di riferire all’Assemblea secondo le date previste. Nella seduta di lunedı, per la quale non efissato l’orario di chiusura, si svolgeranno le relazioni, le votazioni su eventuali questioni incidentali e tutta la discussione generale. Le repliche e il prosieguo dell’esame avranno luogo a partire dalla seduta antimeridiana dı martedı15 febbraio, anticipata alle ore 9,30. Il termine per la presentazione degli emendamenti e nuovamente fissato per le ore 19 di venerdı11 febbraio. Le altre sedute della prossima settimana restano stabilite secondo il calendario gia approvato.

la risposta del Governo a diverse interrogazioni parlamentari che ho presentato sulla gestione del gruppo Delta-Cassa di risparmio di San Marino. davvero tante: ne ricordo una in particolare, la 4-01884 del 31 luglio 2009. Perche´ io leggo oggi sui quotidiani,

signora Presidente, colleghi, la questione del gruppo Delta e una vergogna: pensiamo a come estato ridotto questo gruppo e a come furono concesse le autorizzazioni, sbianchettando addirittura le delibere dalla Banca d’Italia. Ripeto, ho presentato ben sette interrogazioni parlamentari, che c’e una sorta di cricca. Il dottor Patalano, l’avvocato Ferro Luzzi, il dottor Santonocito, il dottor Papi, il dottor Caringi, il dottor Loperfido: tutti uomini che fanno riferimento alla Banca d’Italia. all’avvocato Michele Desario, figlio di Vincenzo Desario, ex direttore generale della Banca d’Italia. Qui che eaccaduto? Che un gruppo e stato commissariato dopo l’inchiesta della procura